nella seduta di *question time* di domani, alle ore 16, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Paolo Gentiloni Silveri, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti:

senatori intervenuti hanno messo in discussione, criticandola chi aspramente e chi in maniera più blanda, la credibilità delle previsioni del Documento di economia e finanza,

e nei primi mesi del 2016. Un po' tutti gli istituti hanno rivisto al ribasso le previsioni di crescita nel mondo, in Europa e, quindi, anche nel nostro Paese. All'altra obiezione secondo cui le nostre previsioni sono ancora troppo alte perché si collocano ai limiti delle verifiche e delle posizioni del consenso - come si dice - credo di poter rispondere dicendo che il Governo

nazionali alla crescita. Del resto, vediamo anche alcuni importanti risultati di questa politica se è vero, come è vero, che viene messo in discussione il calcolo della crescita potenziale

ad esempio - alla riforma della pubblica amministrazione. Qualcuno ha chiesto se le partecipate verranno riformate: la risposta sta proprio nell'attuare la riforma della pubblica amministrazione. Così come, per quanto riguarda gli investimenti,

la parte italiana del piano Juncker, che prevede una leva di 12 miliardi di investimenti da realizzare nel corso del 2016. E, per quanto riguarda il Mezzogiorno più volte citato, c'è tutto il tema del*masterplan*, dei fondi europei

che sono state accompagnate da molti dubbi nel corso degli interventi, noi possiamo rispondere, in modo oggettivo, che le riforme poste in essere, quelle già approvate e da attuare e gli obiettivi programmatici del DEF contengono questa impostazione molto seria, seria, per quanto riguarda sia il controllo della spesa - come si rivela anche dagli indici e dalle previsioni programmatiche - che il sostegno attivo alle politiche per gli investimenti, che si accompagnano alle politiche per il lavoro e alla riduzione della tassazione a vari livelli per

n. 100, relativa alla relazione al Parlamento, con la quale il Governo ha chiesto l'autorizzazione a una modifica del piano di rientro. Riprenderò questo argomento successivamente, ma intanto formulo il parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 100.

presentata dai senatori Uras e Stefano, vorrei svolgere qualche considerazione ulteriore. Il Governo è orientato ad assumere sul piano politico gli impegni previsti in questa risoluzione, facendo presente in particolare di aver già compiuto nella direzione sollecitata scelte precise nel corso degli ultimi due anni. Ricordo il credito d'imposta automatico per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla legge di stabilità per il 2016, la fiscalizzazione degli oneri contributivi per i neoassunti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno anche per il 2017, gli interventi di risanamento ambientale come nel caso della cosiddetta terra dei fuochi. Ma il Governo, sia pur richiamando il senso di tali scelte, riconosce l'urgenza di collocare queste stesse scelte e altre che sta per compiere, e soprattutto i patti per lo sviluppo realizzati e da realizzare con le Regioni del Sud, in un disegno strategico più ampio che utilizzi appieno le potenzialità del Mezzogiorno in termini di risorse umane, territoriali, culturali e ambientali. Ragioni tecniche legate alla specificità della funzione delle risoluzioni sul Documento di economia e finanza, che - come è noto - debbono fissare i confini finanziari e gli obiettivi della sessione di bilancio, impediscono al Governo di trasformare trasformare il consenso politico in un parere favorevole su questa risoluzione. Invito pertanto al suo ritiro per evitare un parere negativo che contraddirebbe - come ho detto - le intenzioni politiche del Governo su questo cruciale tema.

in larga misura condivisibili - lo dico ai senatori che l'hanno proposta - le proposte di impegno indicate in questa risoluzione, specie là dove essa indica chiaramente il collegamento tra riforme dell'assetto politico costituzionale e riforme strutturali per il rilancio dell'economia a partire dal Mezzogiorno. Si tratta peraltro di impegni largamente ricompresi nella proposta di risoluzione n. 5, che il Governo ha poco fa accettato. Per le ragioni tecniche già richiamate, a proposito della specifica funzione delle risoluzioni parlamentari parlamentari sul Documento di economia e finanza, il Governo, che deve accettare una sola risoluzione sul DEF, così da renderla emendabile,

Signor Presidente, dopo la formulazione dei pareri sulle risoluzioni presentate, mi consentirà di svolgere rapidamente alcune considerazioni sui temi di discussione di carattere politico più generale, relativa a questo Documento di economia e finanza. Il tema più ricorrente nella nostra discussione è stato certamente quello della La senatrice Zanoni e il relatore Santini hanno già fatto notare come in verità

dell'autorevolezza rafforzata dalle nomine effettuate dal Parlamento, dai Presidenti di Camera e Senato, circa la direzione di quell'Ufficio e della indipendenza necessaria per fare valutazioni attendibili delle previsioni. deriva, signor Presidente, signori senatori - per chi è interessato all'argomento - un continuo processo di avvicinamento tra previsioni e dati della realtà. Sul prodotto interno lordo - per esempio - si è passati dall'errore medio del 2 per cento tra previsioni e andamento reale *performance* realizzata dall'ultimo Governo Berlusconi) all'1,3 per cento del Governo Monti (sempre in termini di scostamento tra previsioni e dati della realtà),

considerare che ci sia un poco di virtù e di determinazione politica anche nel risultato positivo da noi ottenuto. Ma il costante avvicinamento

quella riforma strutturale che abbiamo introdotto con la presenza dell'Ufficio parlamentare del bilancio nelle stesse procedure di bilancio sta determinando frutti importanti, perché la decisione di bilancio viene fondata su previsioni più attendibili e non perché la qualità del Governo è migliore. Io penso anche che sia così - mi consentirete questa vanità essendo parte del Governo - ma ritengo che ci sia dietro un fatto strutturale e istituzionale che forse, essendo frutto del lavoro di tutti, potrebbe essere da tutti rivendicato. Una seconda osservazione vorrei fare in relazione

per la quale il Governo ha chiesto al Parlamento esplicita autorizzazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, cosiddetta rafforzata, attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione. Mi riferisco di modificare il piano di rientro precedentemente definito per un complesso di fattori che motivano questa proposta del Governo e spero l'accettazione della richiesta di autorizzazione da parte del Parlamento.

Noi pensiamo che la nostra scelta derivi direttamente e sia motivata dall'insufficiente coordinamento delle politiche fiscali ed economiche nell'area dell'euro, in cui politiche di bilancio eccessivamente restrittive potrebbero aggravare le già forti tendenze di tipo deflazionistico e, quindi, forti tendenze alla stagnazione economica. In particolare, su questo punto vorrei aggiungere che è molto al di sotto delle esigenze la politica di espansione dei consumi e degli investimenti nei Paesi in *surplus* eccessivo, non in *surplus* commerciale, ma in eccessivo *surplus* commerciale, secondo le regole europee e non secondo il parere di Enrico Morando. poi incompleta - è il secondo punto - l'architettura dell'Unione bancaria, perché manca la garanzia europea sui depositi. Questo è il primo fattore rilevante su cui voglio richiamare l'attenzione: se non si produce una svolta nel coordinamento delle politiche fiscali,

i Paesi in clamoroso *deficit* e disavanzo di bilancia commerciale faticano a realizzare le riforme strutturali necessarie (penso alla Grecia) che li rendano più competitivi. È dentro questo squilibrio che già c'è la crisi drammatica dell'area dell'euro nella sua capacità di dotarsi di una politica fiscale che risulti efficace nell'affrontare gli *shock* asimmetrici che, in presenza di questa distanza, naturalmente hanno effetti particolarmente negativi. secondo fattore rilevante è la non piena assunzione, nelle regole per il coordinamento della politica fiscale, delle conclusioni a cui è giunta la letteratura economica circa la dimensione del moltiplicatore delle politiche fiscali durante e dopo una profonda recessione. Ormai le analisi anche ufficiali, condotte - per esempio - dal Fondo monetario internazionale, sono chiare: quando un Paese conosce o ha conosciuto una recessione profonda (è il caso dell'Italia), il moltiplicatore delle politiche fiscali, cioè l'effetto di politiche restrittive di bilancio sul prodotto, è molto più grande che in situazione di equilibrio economico. Se si continua ad agire per migliorare le regole di coordinamento e per la sorveglianza sui bilanci senza considerare questo fondamentale elemento, che non è un argomento di tipo tecnico, ma è un fondamentale argomento di orientamento di politica economica e fiscale, non raggiungeremo gli obiettivi che ci prefiggiamo. Da questo punto di vista, quindi, siamo in presenza di un contesto nel quale il coordinamento delle politiche fiscali alla dimensione europea è troppo lontano dalle esigenze proprio sul punto che riguarda riguarda la determinazione delle regole funzionali alla capacità di affrontare e risolvere squilibri eccessivi che si manifestano all'interno dell'area dell'euro. Anche per questa ragione - mi rivolgo in particolare alle forze di opposizione, le quali legittimamente contrastano il Documento di economia e finanza - mi aspetto invece che, sulla richiesta di autorizzazione a cambiare il ritmo e il carattere del piano di rientro, proprio queste forze, che ci sollecitano continuamente ad agire

rimandando per il resto alla replica che ho svolto in Commissione bilancio, che ovviamente, com'è possibile in quella sede, è stata più analitica - un altro tema molto richiamato negli interventi è il livello della pressione fiscale, in particolare sui produttori, e cioè lavoratori Quando questo Governo ha iniziato a operare due anni fa, lo specifico livello della pressione fiscale sulle imprese era ai vertici della graduatoria europea. Se non avete intenzione di prestare fede a quanto dico, andate a consultare il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica per il 2014

tra tutti i Paesi europei. A distanza di due anni, oggi - nemmeno a farlo apposta - c'è stata la pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi al prelievo fiscale sulle imprese nel biennio 2015‑2016. Per gli amanti delle espressioni tecnicamente corrette, il misuratore della pressione fiscale sulle imprese si chiama *total tax rate* ed è un indice di pressione specifico relativo alle imprese, per il 2016 - cito il comunicato di oggi dell'ISTAT - l'effetto complessivo dei provvedimenti assunti è una diminuzione cento delle imposte sulle imprese per un importo pari a 3,5 miliardi. È un risultato impressionante che dovrebbe essere rivendicato come un risultato dell'intera comunità nazionale, perché la riduzione della pressione fiscale sull'impresa, cioè del *total tax rate*, è un obiettivo che anche in passato i Governi si sono proposti senza riuscire minimamente a conseguirlo. Ciò vuol dire che su questo punto siamo arrivati dove vogliamo? No. No. Abbiamo fatto un passo nella direzione giusta, ma vogliamo arrivare al 2018 a un livello di pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro in Italia analogo a quello in vigore in Germania. Perché parlo di Germania? La cito perché è la prima manifattura d'Europa e noi siamo la seconda. Se ogni giorno i lavoratori e le imprese italiane cominciano la competizione con i principali competitori tedeschi gravati da un livello di pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa

là. Perché è importante sottolineare il risultato che oggi viene certificato? Quel risultato dimostra che possiamo farcela. Se in due anni abbiamo ridotto il livello di pressione fiscale sulle imprese mediamente dell'11 cento, significa che la riduzione di ulteriori dieci punti, che ci consentirebbe di arrivare al livello di *total tax rate* della Germania, è nelle nostre possibilità. Basta volerlo con determinazione - e il Governo lo vuole con determinazione - ed essere coerenti, soprattutto sulle scelte di revisione della spesa pubblica che sono essenziali per rendere credibili obiettivi di riduzione della pressione fiscale come quelli che ci proponiamo. *(Applausi dal

Signor Presidente, considerato che il Governo ha dichiarato un sostanziale orientamento ad assumere nel piano politico gli impegni che noi prevediamo nella nostra risoluzione,

in sofferenza. Il Mezzogiorno e le isole lo sono senz'altro. Il Vice Ministro ha fatto riferimento anche ad alcuni provvedimenti che il Governo ha adottato in questi anni, che noi evidentemente consideriamo insufficienti a raggiungere gli obiettivi posti nella nostra risoluzione, ma guardiamo di buon grado a questa apertura e, quindi, all'assunzione di un impegno politico.

Signor Presidente, ringrazio anzitutto il vice ministro Morando per la sua replica, che non ci ha lesinato di osservazioni

ancora una volta una pericolosa dissociazione tra ipotesi e realtà a danno di cittadini, famiglie e imprese, a partire dai dati su crescita e inflazione. Vice ministro Morando, la sequenza storica che lei ha citato sui dati discostanti tra previsioni e realtà non ci consola a sufficienza. è solo con un significativo incremento del prodotto nominale che è possibile rimanere nei parametri europei del *deficit*, e soprattutto - dico io - del debito, la cui riduzione, prevista già enfaticamente per quest'anno, è per il Governo un obiettivo strategico, ma intanto rinviato. A tale riguardo ricordo che, lo scorso anno, lo *stock* di debito è aumentato di 35 miliardi, che valgono oltre due punti di PIL; la stima del rapporto per il 2016 è stata rivista in peggio di un punto percentuale (un punto percentuale e non lo 0,2), ovvero circa 17 miliardi, rispetto a quella recente di settembre, contenuta nella Nota di variazione al DEF 2015, frutto in buona parte - come lei sa, Vice Ministro - del peggioramento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni; che la previsione per il 2016 sconta l'apporto positivo delle privatizzazioni per circa 8 miliardi: una una cifra tutta da verificare, per come si sono messe in moto le privatizzazioni nel nostro Paese, soprattutto insieme alle modalità di realizzazione. Insomma, se il rischio che le stime programmatiche siano meno buone del previsto è molto fondato, quanto è sostanziale la sostenibilità di un debito che, in valore assoluto, continua a crescere significativamente anno dopo anno? L'aumento del debito è un dato preoccupante - lo abbiamo sempre segnalato, vice ministro Morando, e non da oggi - frutto del ricorso sistematico da parte del Governo al *deficit* come strumento per preservare politiche fiscali cosiddette espansive, invece che attuare una vera riduzione della spesa pubblica, quella sì realmente espansiva. Ma la critica al DEF 2016 potrebbe continuare su molti altri aspetti.

Il Governo ritiene che la crescita si ottenga solo agendo dal lato della domanda - e questo è un dibattito al quale da tempo partecipiamo ampliandola però con il ricorso al *deficit* e a specifiche misure di stimolo che spesso, però, si rivelano frammentarie, a volte denominate anche mance o regalie, con effetti pressoché inutili allo scopo. Questa è la dimostrazione di come gli 80 euro, che potrebbero diventare 100, che hanno avuto e avranno il minimo pregio di accontentare qualcuno - contro un pesantissimo aggravio per la collettività - non daranno certamente i frutti sperati dal Governo.

impedisce di far fronte a impieghi protratti nel tempo con risorse denominate e definite a breve, pena la non sostenibilità di quegli impieghi e il fallimento dell'azienda (ma l'azienda è il nostro Paese e a fallire rischiamo di essere tutti noi). raccontare in tutte le occasioni che la crescita - quella che noi non vediamo - del nostro prodotto è dovuta ai consumi, agli effetti di misure come i famigerati 80 euro (e ai conseguent*i deficit* conseguiti per la loro attuazione) ha come come risultato un bel titolo sui giornali e nessun cambiamento nella vita quotidiana delle persone e delle famiglie, oltre che far perdurare una situazione di emergenza continua. Insomma, sembrano belle parole, ma poi le cifre sono bruttissime. Certo, la domanda ha un suo ruolo nello sviluppo, ma oggi più che mai, per una crescita robusta e duratura, è necessario agire sull'offerta, con strumenti che non operano necessariamente nel breve periodo e che incrementano la produttività, altro fattore critico della nostra economia, che ci vede in fondo alle classifiche europee. Servirebbe, secondo noi - e ne siamo sempre stati convinti - oltre che ridurre spesa pubblica, un coraggioso piano di investimenti veri nelle infrastrutture materiali e immateriali del Paese, che abbiano ricadute vantaggiose per tutta la collettività, soprattutto utilizzando quella leva fiscale che invece non si vuole mai usare. Non sarebbe arrivato il momento, ad esempio, di portare l'alta velocità nel Sud? Non sarebbe necessario realizzare reti e infrastrutture energetiche che nel Nord del Paese, come nel Sud, rendano possibile rendano possibile cogliere le opportunità derivanti, ad esempio, dalle importanti scoperte di giacimenti di gas naturale nel bacino del Mediterraneo, permettendo, nel contempo, il graduale calo del costo dell'energia, a vantaggio di imprese e consumatori, con rilevante contributo all'abbattimento delle emissioni inquinanti? Da questo punto di vista, oltre all'enfatico proclama di una ripartenza degli investimenti sin dal prossimo anno, nel Documento si fa riferimento solo al piano Juncker, che io apprezzo molto, ma che stenta a decollare, mostrando limiti ed ambiguità operative. Ora più che mai ci sarebbe bisogno di interventi veri per il mercato del lavoro, non quelli paradirigistici del *jobs act*, che ha portato striminziti vantaggi a fronte di enormi costi pubblici. Piuttosto, quelli che puntano ad una liberalizzazione effettiva del mercato, ai contratti aziendali piuttosto che al *moloch* del contratto collettivo nazionale del lavoro, quello che contiene ancora misure molto rigide all'interno del mercato del lavoro; misure che aiutino l'occupazione. Tutti noi - Governo, maggioranza e opposizione - siamo ovviamente molto attenti al tasso di disoccupazione, ma spesso dimentichiamo quello di occupazione, che nell'ultimo decennio è in costante discesa. Le misure attuate dal Governo negli ultimi anni non sembrano andare nella direzione auspicata: penso ai risultati deludenti della cosiddetta «garanzia giovani» o a quelli degli sgravi Abbiamo bisogno di lavorare di più e molti di più devono lavorare se vogliamo rendere sostenibile il nostro sistema pensionistico, che peraltro dimostra di essere sempre più fragile e bisognoso di essere rinnovato profondamente. Servirebbe un coraggioso cambio di marcia per individuare forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria, verso schemi previdenziali integrativi, in particolare a favore delle giovani generazioni, ma non solo. Occorre costruire per i nuovi assunti un trattamento di base, Il ministro Padoan ribadisce l'intento di perseguire una politica una politica fiscale rigorosa e, al tempo stesso, espansiva. Ma è inutile rivedere aliquote o agevolazioni se questo significa maggiore *deficit*. Così continueremo solo a cambiare gli addendi, ma non la somma. È ormai indispensabile rivedere completamente la tassazione su persone e imprese, nel solco di una significativa riduzione delle aliquote e, con riferimento all'imposizione personale, di un sostegno alla famiglia, anche mediante l'introduzione di meccanismi come l'*income splitting*, che riducono la progressività e il carico fiscale

Mi compiaccio, vice ministro Morando, per la sua citazione del *total tax rate*: quella è la strada da seguire e mi auguro che ci si possa arrivare il più velocemente possibile. Una revisione, quella delle *tax expenditure*, che dovrebbe tenere conto delle scelte di innovazione, di ristrutturazione e di aggregazione adottate dalle imprese, dalle quelle micro a quelle piccole e medie, dobbiamo sostenere soprattutto nell'accesso al credito. Credito e sistema bancario non possono essere esposti, anche a causa della debole azione di questo Governo, come di quelli che lo hanno preceduto, allo scontro con la visione sbagliata, tutta europea, anzi, per meglio dire tutta tedesca, tutta tedesca, che stiamo subendo da troppi anni. Le procedure di ricapitalizzazione, quelle interne previste dalla direttiva comunitaria, tra cui il famigerato *bail in,* vanno riviste, per non scoraggiare i cittadini ad impiegare il proprio risparmio nelle imprese bancarie, evitando rischi concreti per la stabilità finanziaria del Paese. Personalmente considero un piccolo buon inizio l'operazione che va sotto il nome di Fondo Atlante e il ruolo svolto dalla Cassa depositi e prestiti fuori dal perimetro del debito pubblico e degli aiuti di Stato. Un'operazione che ci mette al riparo da rischi molto impellenti, fatta dal sistema per il sistema. Ciò non toglie che questo DEF non solo delude noi, ma deluderà anche gli italiani, ancora una volta. Signor Presidente, mi permetta di iniziare con una lamentela sui tempi della discussione sul DEF.

per poterle evitare: 15 nel 2016, 20 nel 2017 e 20 nel 2018. Il dubbio è: ma come farà?

E questo cosa comporta? Che tutti siamo qua a vivere un'incertezza. Vivranno l'incertezza i Comuni e le Regioni, perché non sanno quale sarà il loro futuro e loro stessi non potranno fare una programmazione, perché basta che il Governo, come abbiamo visto recentemente, applichi dei tagli e un Comune che magari ha fatto una previsione

Poi però cita: il Governo cosa vuol fare? Razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale e previdenziale, introducendo il principio di universalismo selettivo.

la diminuzione della spesa, anche qua è facile dirlo. Però a spese di chi? Non certo dei Ministeri e del Governo centrale, ma a spese dei Comuni e delle Regioni; ci sono tutte le tabelle che lo dimostrano. C'è il problema del *turnover* dei Comuni; a causa

Senza contare il fatto che la rivoluzione del sistema bancario non è a favore dei cittadini, ma forse a favore solo dei grandi banchieri. Un'ultima riflessione riguarda il tema della sicurezza, che è un tema importantissimo e fondamentale. Un cittadino si deve sentire sicuro a casa

MPL))*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, care colleghe e colleghi, ci sono dei giorni - e questo è uno di quelli - in cui

sbandierato come grandi successi, grandi aspettative o grandi programmi di cambiamento fanno i conti con i dati, con i numeri e con la realtà. Per criticare il DEF che è sottoposto alla nostra attenzione non mi servirò delle argomentazioni o dei riferimenti numerici di questa o di quell'altra parte politica, ma utilizzerò gli stessi strumenti, le stesse parole e le stesse relazioni che appena due anni fa ha svolto e ha

questo Governo nell'anno 2014, rispetto a cosa scrive oggi il Governo, nell'anno 2016, nella propria relazione. prende atto di non aver centrato nessuno degli obiettivi che si era proposto appena due anni fa. Prende atto del fatto che la crescita, l'abbassamento dell'indebitamento, la realizzazione dei livelli occupazionali, tutti i dati e tutti i riferimenti macroeconomici, ma anche quelli relativi all'economia reale, sono tutti

l'ammissione di una incapacità a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma trovo scandaloso che un Documento importante e fondamentale, che da un lato deve fotografare la situazione del Paese e dall'altro deve porre le basi fondamentali della futura legge di stabilità per l'anno 2017, sia così sterile dal punto di vista della capacità progettuale e della capacità di indicare la strada per l'uscita dalla crisi.

a non fotografare un'Italia con delle difficoltà gravissime? Perché il fatto che voi nascondiate sotto il tappeto le difficoltà significa che non ponete come base della futura legge di stabilità i problemi reali. E come fare a non preoccuparsi oggi

della maggior parte dei cittadini italiani che vivono al di sotto di Roma? Con quale speranza e fiducia possono vivere i cittadini se noi stessi siamo deprivati della fiducia nei vostri confronti? Utilizzo questa aggettivazione perché mi serve per introdurre un concetto, vice ministro Morando. Lo SVIMEZ, che non è esattamente il centro studi di Forza Italia, ma un organismo che studia i fenomeni, l'economia e l'interconnessione tra gli strumenti di Governo e le esigenze dei territori, utilizza due termini fondamentali: il primo è quello della deprivazione. Vice ministro Morando, la deprivazione è l'indice con cui si individua la povertà delle famiglie,

il vivere sotto il livello della soglia della povertà. Lei di questo indice ne deve parlare, perché un Governo non può non preoccuparsi di come

dal punto di vista sociale è un aspetto che il suo Governo non può minimamente disconoscere e non può farlo certamente la sua maggioranza parlamentare. Che cosa dire poi dall'altra aggettivazione, la desertificazione del Mezzogiorno d'Italia? Un organismo che studia l'economia, che ha a disposizione tutti i vocaboli che vuole nel campo dell'economia,

Sono davvero sconcertato dal fatto che ancora una volta si vengono a ripetere i soliti ritornelli: si parla ancora dell'intervento nel Mezzogiorno attraverso la defiscalizzazione del lavoro. Lo volete capire che nel Mezzogiorno il lavoro non c'è? Se c'è qualcuno che si premura di definire desertificato quel territorio, il problema è proprio quello di creare la produzione, i processi

alla possibilità di spesa dei fondi della programmazione comunitaria 2014-2020. la tranquillità e la fiducia che ispira un testo nei confronti di un problema che ha caratteri così profondi, che genera condizioni così strazianti dal punto di vista sociale ed economico?

l'Italia non raggiungerà quei livelli di PIL che le potranno consentire di pagare il debito pregresso se non affronterà e recupererà la capacità di crescita del PIL e dell'economia complessiva nel Mezzogiorno d'Italia.

ad inserire nel DEF 2016 l'adozione di un Piano straordinario per il Mezzogiorno che abbia una visione di insieme e di durata; Io ritengo che sia sufficiente per il Governo, per l'Assemblea in generale e per il senatore Mauro che proprio su questo punto porremo una condizione politicamente corretta, ma molto incisiva. preso qualche appunto, ma lo spunto che mi ha dato il Governo è molto interessante,

relativamente a una questione di carattere generale. Noi abbiamo condiviso e condividiamo che ci sono delle priorità parlo di politica di bilancio - e tra le priorità vi è la riduzione del carico fiscale e la ripresa degli investimenti. È da lì che vogliamo sviluppare il nostro ragionamento per aiutare il Paese nel suo complesso, per dichiarare - lo dico molto convintamente - che le riforme avviate, sia quella della pubblica amministrazione che la riforma sul lavoro, vanno nella giusta direzione.

di decisioni che vengono prese solo da una parte. L'accavallarsi di sovrapposizioni non fa altro che paralizzare tanto il sistema amministrativo quanto il mercato. Tutto

dai Comuni, alle Regioni, alle ex Province (ancora non si capisce in alcune Regioni dove si va a finire), dove non c'è mai una decisione vera, o comunque una vera decisione.

Perché noi no e nelle altre aree del mondo sì? Poniamocelo questo interrogativo, perché il Paese ha bisogno di essere integrato, interconnesso. Non è più ammissibile - lo dico perché ne è a conoscenza il Governo certamente prima di me per andare da Bari a Reggio Calabria occorrano otto ore e magari per andare da Bari a Milano se ne impieghino tre

che è ancora più scandaloso e vergognoso, perché non ci sono né porti, né aeroporti, né strade, né ferrovie.

citare coloro i quali ci hanno preceduto nei secoli, nell'ultimo cinquantennio, che hanno tentato di mettere mano al Mezzogiorno. Ma oggi ci sono tutte le condizioni

Io da siciliano sono a favore del ponte, ma dopo aver ultimato le priorità come le infrastrutture primarie, le strade le autostrade. Ci sono circa 20 chilometri per chiudere l'anello circoscritto. Parlo, per ora, della Sicilia.

completamente dal sistema Paese. Questo lo abbiamo detto e lo ribadiamo soprattutto per le opere incompiute, signor Vice Ministro.

e importanti che servono al Paese. Basta fare le sagre della salsiccia con i fondi europei. Assumiamoci la responsabilità. La sagra delle salsicce se le facciano i sindaci e i Comuni.

Saldare il Paese significa fare una grande scommessa. Ribadisco ancora: oggi ci sono tutte le condizioni. Un euro

utilizzi questa equazione anche per il Mezzogiorno: un euro speso per il Mezzogiorno, un euro speso per la cultura.

il 2017 e per il 2018, possono essere importanti per il Mezzogiorno e per il Paese. Noi ci crediamo fortemente

che stanno assistendo ai nostri lavori. Signor Presidente, colleghi, lo sforzo del Governo in questi anni poteva essere sicuramente profuso meglio, più ampio e più incisivo, al fine di produrre risultati più significativi. È vero, c'è stata in questi ultimi due anni una minima crescita economica e un incremento - anche questo minimo - dell'occupazione. Il Governo, però, avrà ancora molto da fare: deve porre maggiore attenzione agli investimenti, sia pubblici che privati, in funzione della previsione di un aumento del prodotto interno lordo

L'impresa più difficile rimane comunque quella di creare lavoro. La disoccupazione è prevista per quest'anno all'11,4 per cento; il 2017 è prevista invece al 10,9 per cento: anche questa si vede scendere di mezzo punto, ma rispetto ai milioni di disoccupati che ci sono la sfida diventa difficile e importante. Le politiche attive del lavoro faticano a prendere il via; non viene fatto abbastanza per valorizzare il nostro capitale umano e soprattutto i nostri giovani, non si è ancora risposto in maniera concreta al problema della flessibilità in uscita verso il lavoro e verso coloro che vogliono andare in pensione. C'è molta strada da fare per cercare di reperire anche il tanto denaro sommerso che gira nel nostro Paese. Occorre, quindi, maggiore controllo, maggiore legalità; arginare l'evasione e la corruzione, recuperare l'IVA, come ricordava anche la senatrice Guerra. Dobbiamo, la senatrice Guerra. Dobbiamo, quindi, diventare un Paese più credibile e affidabile agli occhi dell'Europa, ma soprattutto per il nostro Paese, per aumentare il nostro benessere e fare in modo che l'ultimo della fila viva dignitosamente; la strada è pertanto in salita.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, la crescita italiana registrata nell'ultimo anno è messa in pericolo da fattori negativi determinati da un contesto internazionale che presenta un insieme di problematiche che influiscono inesorabilmente anche sul nostro Paese, e non solo sulla sua crescita economica ma anche sulla sua sicurezza. Questo ha determinato la revisione al ribasso delle stime di crescita rispetto alla Nota di aggiornamento dello scorso autunno e un più graduale piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine. A questi fattori si aggiungono - come abbiamo avuto modo e occasione di discutere, anche insieme al Vice Ministro, in Commissione - anche le criticità emerse in relazione alla metodologia adottata dalla Commissione europea per il calcolo della crescita potenziale e dell'*output gap* alla base della stima del saldo strutturale di finanza pubblica. Tale metodologia - è opportuno ribadirlo in quest'Aula - come più volte sostenuto anche dal Governo e come riportato nello stesso DEF, fornisce risultati sottostimati, che si scostano rispetto ad altre metodologie di calcolo quali quelle seguite dall'OCSE, con la conseguenza che con quest'ultima metodologia, a differenza dell'altra, avremmo raggiunto già nel 2015 l'obiettivo di medio termine. Gli obiettivi che il Documento si propone sono quindi fortemente condizionati da questi fattori e da quanto avviene fuori dai nostri confini, imponendo una riflessione a più ampio raggio. Fenomeni come quelli della pressione migratoria stanno creando enormi problemi e stanno mettendo in crisi la stessa coesione europea e il recente voto in Austria è la dimostrazione di questo dato. Le notizie che, peraltro, oggi arrivano dal Brennero sono alquanto allarmanti:

Il nostro Paese, per la sua posizione geografica, è infatti uno dei Paesi più esposti a questo flusso migratorio, ma è anche quello che ha una più forte cultura dell'accoglienza. L'Europa si è dimostrata e si sta dimostrando impreparata e rischia di frantumarsi a causa delle iniziative politiche che stanno adottando i singoli Stati dell'Unione, che manifestano una forte preoccupazione per il ad adottare azioni di contrasto contrarie allo spirito di unità e solidarietà che dovrebbero invece animare l'Unione europea. Difficoltà che sono aggravate dalle difficoltà economiche generali, ad esempio dal rischio di una futura uscita - a breve futura uscita - a breve - da parte della stessa Gran Bretagna dall'Unione oppure dalla questione greca che è riesplosa in questi giorni. Sono quindi sempre più evidenti i limiti di questa istituzione, che non riesce a superare le spinte nazionaliste che si riaffacciano regolarmente nei momenti di difficoltà. Una istituzione che non ha di fatto i poteri necessari per contrastare le situazioni di crisi quando si presentano, anche a causa di una diversità di culture di governo, mentre oggi sarebbe quanto mai auspicabile una politica comune europea in settori strategici, quali la politica estera, la politica economica e fiscale dell'Unione. Gli sforzi che il nostro Governo sta compiendo in questo senso sono estremamente utili e fondamentali e devono essere supportati. Occorrerebbe, in particolare per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari, un Ministero unico o comunque un coordinamento delle politiche fiscali - come ha ribadito poco fa lo stesso Vice Ministro in questa sede - la cui assenza rappresenta un grave *handicap* per l'eurozona. Dal documento al nostro esame traspare così una certa cautela

Il calo dell'*export* e il conseguente calo della produzione nel nostro Paese è legato anche al rallentamento delle grandi economie emergenti. Anche se non ci troviamo di fronte alla fase acuta della crisi iniziata nel lontano 2008 queste difficoltà pesano sull'Europa, che ha rallentato il suo processo di crescita crescita appena avviato e che nei mesi scorsi aveva fatto ben sperare, vanificando in parte anche gli sforzi compiuti dalla BCE attraverso la leva monetaria. Un Paese come l'Italia che ha un debito pubblico elevato

Dobbiamo quindi riconoscere che rispetto a tutte queste situazioni di incertezza il Governo e il Parlamento stanno facendo la loro parte. In particolare, c'è l'impegno del Governo a sterilizzare nella prossima manovra di bilancio le clausole di salvaguardia mediante l'utilizzo degli spazi di flessibilità richiesti. Diversi sono stati i provvedimenti di svolta rispetto al passato approvati. Il processo riformatore, che con tanta caparbietà si sta portando avanti e i cui effetti si vedranno nel tempo, è un processo che ha dei costi, non solo ovviamente in termini economici ma anche in A questo proposito riteniamo che, per dare un fattivo contributo a quanto si sta compiendo anche in questi mesi per assicurare al nostro Paese un futuro migliore, sia necessaria un'efficace azione culturale. Ci stiamo riprendendo, ma le aspettative sono ancora molte, forse troppe, tuttavia nessun Governo in un'economia globalizzata può dirsi immune, tantomeno il nostro che non possiede la bacchetta magica e che ovviamente non può annullare le influenze negative esterne. Da qui l'esigenza di alimentare maggiormente la ripresa economica con politiche di stimolo e il DEF 2016 si inserisce perfettamente nella strategia di programmazione economica pluriennale intrapresa, che ha come obiettivi principali il rilancio della crescita e dell'occupazione. Dopo due anni di Governo è possibile fare un primo bilancio. Alla base di questa politica ci sono le riforme istituzionali, che hanno lo scopo di consentire una maggiore stabilità politica, premessa per l'assunzione di provvedimenti che avranno i loro effetti nel medio e lungo termine. In questo senso, il Parlamento e il Governo hanno già approvato una serie di provvedimenti intesi, tra l'altro, a semplificare la struttura della pubblica amministrazione. Questa è una riforma che riteniamo fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la rivisitazione della spesa. Una leva importante è l'impegno a sbloccare le opere pubbliche, anche attraverso la revisione delle modalità di assegnazione degli appalti, che richiedono maggiore trasparenza e soprattutto controlli, per evitare i fenomeni corruttivi che purtroppo affliggono ancora il nostro Paese. Condivisibile è pertanto la stima conservativa adottata dal Governo sulla crescita per il 2016, affidando la prospettiva di miglioramento al triennio successivo in considerazione degli interventi previsti. Importante sarà lo stimolo agli investimenti che il Governo riuscirà a realizzare pur in presenza di un contesto economico internazionale incerto. Molto si è fatto in questi ultimi anni e, da ultimo, con la legge di stabilità per il 2016 e molto si dovrà fare, sopratutto per favorire gli investimenti esteri. Gli interventi approvati in questi anni stanno offrendo i primi risultati. Certo, non come quelli che si aspettavano in termini di abbassamento del tasso di disoccupazione, però anche questo testimonia che vi è una rinnovata fiducia e una parziale ripresa degli investimenti pubblici e privati. L'indice della pressione fiscale segna una diminuzione che lascia ben sperare per il futuro e per la politica di riduzione della pressione fiscale stessa, che il Governo ha intenzione di attuare sia nei confronti dei cittadini, che delle imprese. Auspichiamo, visti i risultati ottenuti in termini di crescita, che la riduzione del cuneo fiscale possa diventare una misura permanente e che nella rivisitazione della redistribuzione fiscale sia prestata particolare attenzione alle fasce più deboli. A questo scopo, un contributo potrà arrivare da una energica politica di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Un tema particolarmente sensibile, sia per ragioni

annuale, insieme alla Nota di aggiornamento al DEF, del Rapporto sui risultati conseguiti in termini di contrasto all'evasione e le nuove strategie programmate. Un contributo importante potrà arrivare anche dall'annunciata fatturazione elettronica tra privati. Ciò consentirà un maggiore controllo sul gettito delle imposte indirette. Importanti saranno anche gli interventi previsti per quanto riguarda la semplificazione della giustizia civile, che è volta ad accelerare anche la dismissione dei crediti in sofferenza da parte delle banche, fattore importantissimo per far ripartire una politica del credito. Le stesse privatizzazioni che sono state programmate per i prossimi anni, per quanto ci sia da essere prudenti nel contesto generale, rientrano chiaramente in una politica di abbassamento del debito che condividiamo. maggiori margini di flessibilità che oggi interessano noi italiani, in futuro potrebbero essere richiesti anche da quei Paesi con un debito pubblico più contenuto. Faccio questa affermazione perché secondo un'autorevole fondazione tedesca, la Stiftung Marktwirtschaft - e lo dico soprattutto alla luce di quanto detto ieri dal presidente della Bundesbank proprio qui in Italia - il debito pubblico totale italiano è l'unico nella Unione europea ad essere, nel lungo termine, il più sostenibile (sotto la soglia del 60 per Per debito pubblico totale si intende non solo quello esplicito, cioè quello che abbiamo ereditato dal passato, ma anche quello implicito, che è dato dagli impegni pensionistici, dai futuri costi della sanità e dai costi sociali legati all'invecchiamento della popolazione. Da questo punto di vista, le riforme fatte negli ultimi anni

Quello che si vuol dire è che probabilmente questa flessibilità rischia di essere chiesta oggi dall'Italia e, in prospettiva, anche da chi oggi pensa di avere le spalle coperte.

Penso, in sintesi, alla riduzione della spesa pubblica (quella buona e non i tagli agli sprechi), al rilancio di un'idea di privatizzazioni, all'aumento nei fatti della pressione fiscale sul ceto medio e sulle classi popolari, al taglio indiscriminato e non distintivo delle tasse alle imprese, al sostegno agli investimenti privati attraverso gli sgravi fiscali e alla precarizzazione del mercato del lavoro. È ormai evidente l'assoluta inefficacia di queste politiche che non sono in grado di promuovere la crescita, creare lavoro stabile e duraturo, ridurre l'enorme debito pubblico e arginare la crescita della povertà e del disagio sociale. la presenza di una strategia di comunicazione molto attenta da parte del Governo e di Renzi a carpire il consenso e gli annunci sulla fine dell'*austerity* e sulla crescita non riescono più a sortire gli effetti di prima, a causa ormai sempre più acclarata assenza di politiche economiche che puntino realmente al superamento della crisi e dell'austerità e finalizzate a uno sviluppo che offra benessere e progresso sociale. Mancano politiche serie dell'occupazione e manca, checché se ne dica continuamente in televisione, una vera e propria politica industriale. presenta, ancor più che in passato, come un contenitore di indicazioni approssimative, disomogenee e contraddittorie da cui emergono fondamentalmente quattro cose, a cominciare dalla costante revisione delle previsioni macroeconomiche, sempre riviste al ribasso

con cui si calcola il Patto di stabilità europeo e la conseguente quantificazione di quanto margine in più di finanza pubblica programmatica si intende chiedere all'Unione europea. Emergono, infine, una lunga lista di effetti sovrastimati delle riforme avviate dal Governo e, infine, una grandissima avarizia su ogni particolare che riguardi le misure di attuazione degli obiettivi contenuti nel DEF, che di regola sono appresi solo all'ultimo momento con la presentazione, in autunno, della Nota di aggiornamento e della legge di stabilità.

in peggioramento, irrealistici ed eccessivamente ottimistici, come quelli sulla disoccupazione. Le risorse deriveranno principalmente da nuovi tagli alla spesa e da tagli previsti alle agevolazioni fiscali. Nonostante la tanto decantata fine dell'austerità, si prevedono quindi nuovi sacrifici e si amplierebbero ulteriormente le misure riguardanti la *spending review* come se, con le precedenti manovre, non avessimo tagliato già 25 miliardi di euro, attuando una manovra che si basa su un *mix* di interventi di revisione della spesa pubblica e di tagli alle agevolazioni fiscali. Proprio su questo tema, tema, vorrei aggiungere i non meglio specificati altri strumenti di contrasto all'evasione ed elusione, che dovrebbero garantire il raggiungimento di un indebitamento netto pari all'1,8 per Ricordiamoci però che la revisione prevista delle agevolazioni, quindi delle *tax expenditure*, si tradurrà di fatto in un altro aumento della pressione fiscale per il ceto medio e per le classi meno classi meno abbienti, trattandosi di tagli a tutte le agevolazioni fiscali sulla casa e sulla famiglia, come le spese per mutui, per la sanità ed altro ancora. La riduzione dell'aliquota IRES prevista dall'ultima legge di stabilità è anch'essa a nostro avviso ingiusta. In un Paese ancora stretto dalla morsa della crisi e con un tasso di disoccupazione oltre l'11 per cento, diminuire in maniera generalizzata un'imposta sui profitti, scelta che, rispetto alle misure su IRAP e decontribuzione che almeno intervenivano sui costi seppur in modo non selettivo, appare un ingiustificato "regalo

nonostante il Governo non si esima dal vantare il *trend* positivo del recupero, pari nel 2015, secondo il Governo, a 14,9 miliardi,

per la riduzione strutturale della stessa la vera chiave di volta per contrastare il debito pubblico ed uscire dal guado. In questo stato di cose l'obiettivo, non più rinviabile per la tenuta della coesione sociale, di ridurre il prelievo fiscale sui redditi di lavoratori e pensionati e di assumere il sostegno alla famiglia come fattore di una maggiore equità distributiva va intrapreso, modificando la composizione del prelievo, compensando il minor gettito con una revisione dei tributi che colpiscono rendite e consumi. Un percorso complementare, che conduca quindi ad una revisione delle modalità di tassazione Il Governo dovrebbe smettere di essere ondivago e dovrebbe affrontare di petto questa situazione.

sgravi fiscali. Nella pubblica amministrazione si vanta la *spending rewiew*, ma in realtà questa è stata sostenuta dalle lavoratrici e dai lavoratori del pubblico impiego. Non a caso, tra il 2009 e il 2015, la spesa per i redditi dei dipendenti pubblici è diminuita di 10 miliardi di euro e il numero dei dipendenti pubblici è calato di 110.000 unità. Per non parlare poi del blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione, che non ha prodotto una razionalizzazione efficace e un miglioramento dei servizi e delle prestazioni.

Inoltre in questo DEF - ne hanno parlato molti - non c'è traccia di politiche per il Mezzogiorno. Il capitolo ricerca, scuola ed università non solo non riserva nessuna particolare sorpresa, ma non fa fa minimamente accenno alla condizione in cui versano attualmente la scuola, l'università e la ricerca pubblica. L'Italia procede nella più grande e sistematica operazione di distruzione del sistema istruzione, università e ricerca, investendo meno dell' 1 per cento del suo PIL in ricerca e sviluppo. Per non parlare poi delle politiche sociali. Io trovo ridicole le politiche che vengono messe in campo per il contrasto alla povertà (ne abbiamo parlato molte volte). A fronte di un aumento di circa un terzo dei cittadini con un reddito al di sotto della soglia di povertà, il Governo propone praticamente di dare un piccolo sollievo a circa 280.000 famiglie, rispetto al milione e mezzo di famiglie che si trovano in una condizione di povertà. alla spesa sanitaria, i dati sono freschi e per la prima volta ci dicono che vi è un calo delle aspettative di vita. Forse dovremo fare una riflessione seria su cosa è la nostra spesa sanitaria in rapporto al PIL, che sta diminuendo sempre di più. Su questo non vi è cenno, come non vi è alcun cenno nel DEF in campo ambientale. I pochi provvedimenti positivi sono stati approvati, ma non sono ascrivibili all'azione di Governo, e potremmo parlarne a lungo. Non vi è niente sulle modifiche e pochissimo sui pendolari, quindi un fallimento di queste politiche che vengono riprodotte nel DEF. Per noi di Sinistra Italiana bisognerebbe cambiare davvero passo e cambiare l'orizzonte delle politiche economiche, abbandonando le politiche di austerità e rimettendo al centro delle scelte un impianto di politiche espansive. Serve un piano straordinario verde del lavoro, così come descritto nella nostra risoluzione; serve affrontare di petto la questione del Mezzogiorno. Noi proponiamo di reintrodurre la cosiddetta clausola Ciampi: un vincolo di destinazione del 45 per cento del totale per investimenti nel Mezzogiorno. Servono inoltre politiche serie sulla scuola, l'università, la ricerca. In campo ambientale abbiamo votato una mozione per la stabilizzazione dell'ecobonus. La direzione è quella: un nuovo piano straordinario energetico e il piano generale dei trasporti. In sintesi, occorre veramente un cambio di passo perché abbiamo avuto tanta propaganda ed esaltazione di riforme che non hanno prodotto risultati dal punto di vista della crescita del Paese. Bisogna assolutamente modificare l'impianto generale delle politiche economiche e puntare, come sul piano straordinario per il lavoro verde, su quelle opere e su quegli investimenti che, come abbiamo già visto, sono gli unici in grado di dare risposte e far crescere seriamente l'occupazione. Per tutti questi motivi, noi voteremo contro il DEF e a favore della nostra risoluzione. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Documento di economia e finanza di quest'anno registra la prima vera inversione di tendenza del nostro Paese dopo la crisi economica degli ultimi anni. Nel 2015 il prodotto interno lordo è aumentato, la disoccupazione e le tasse sono diminuite, e le riforme strutturali per il Paese sono in corso di approvazione e di attuazione. In altre parole, l'Italia si è rimessa in moto ed è tornata finalmente a crescere. Quello che è stato fatto finora ha rappresentato una fondamentale inversione di tendenza, ma allo stesso tempo non può essere che il primo di una serie di punti positivi per una piena e consolidata ripresa. Siamo soddisfatti delle riforme fin qui attuate, dei provvedimenti di rilancio dell'occupazione e degli investimenti. Ma tutto ciò non può che essere uno stimolo affinché Parlamento e Governo continuino sul percorso riformatore. Lungi dal farci sentire appagati, l'anno passato deve costituire la base per uno sviluppo più solido e strutturato, che coinvolga tutti i settori del Paese. La maggioranza e il Governo sono ben consci che gli ostacoli da superare per arrivare ad una piena ripresa sono ancora molteplici e radicati da troppo tempo nel nostro sistema Paese. Le audizioni degli attori istituzionali e industriali tenute dalle Commissioni parlamentari lo hanno dimostrato: le stime macroeconomiche del Governo, se appaiono realistiche e condivisibili, devono mettere in conto dei rischi di potenziali andamenti meno favorevoli, soprattutto a causa di un quadro internazionale, geopolitico ed economico, instabile. La zona euro, nonostante segnali incoraggianti e positivi, non ha mostrato una tendenza tale da scongiurare una prolungata fase di stagnazione e deflazione. Proprio prendendo in considerazione tutte queste variabili, il DEF 2016 ha tracciato un percorso futuro che unisce un nuovo approccio di reperimento delle risorse a modalità di spesa che moltiplichino le capacità di crescita. Le clausole di salvaguardia per il 2017 dovranno essere disinnescate e non ne verranno poste di nuove a garanzia dei conti pubblici. È importante agire, come esposto nel DEF, con un'azione mirata e strutturale di *spending review* e adottando un approccio espansivo rispetto alla rigida disciplina di bilancio prevista dall'Europa. Le risorse così ottenute saranno utilizzate per finanziare una nuova diminuzione del carico fiscale e per garantire gradualmente il rientro all'interno dei parametri macroeconomici concordati con l'Europa, *in primis* il progressivo abbattimento del debito pubblico. È proprio l'ingente debito pubblico il fattore che più deve attirare l'attenzione del Governo e del Parlamento: infatti, la riduzione del rapporto debito/PIL è diventato un obiettivo strategico della politica economica degli ultimi due anni. nel 2015 ha continuato a crescere, seppur leggermente, il 2016 dovrà essere l'anno in cui il debito inizierà la sua discesa, soprattutto in considerazione del fatto che i bassi tassi di interesse di cui l'Italia ha potuto beneficiare negli ultimi mesi non possono durare ancora per molto. È stato giustamente sottolineato, comunque, come tale riduzione dovrà procedere in modo più celere e deciso perché il nostro Paese e anzi attragga, nuovo credito dai mercati e allontani ancora di più i rischi di esposizione a crisi di sfiducia ed eventuali attacchi speculativi. Il nuovo clima di fiducia nelle nostre istituzioni economiche e politiche è alimentato dalla ripresa dell'occupazione e dal miglioramento del potere d'acquisto delle famiglie. Proprio queste ultime sono i nuclei fondamentali da sostenere nella ricostruzione del tessuto sociale: sono stati già adottati provvedimenti importanti nel settore, quali il *bonus* bebè e la carta famiglia. Tali strumenti, positivamente sperimentati, devono essere perfezionati e potenziati, ad esempio modificando i parametri per l'accesso al *bonus* bebè per estendere la platea dei potenziali beneficiari. Visti i dati demografici relativi alla natalità e all'invecchiamento della popolazione italiana, sembra opportuno elaborare nuove politiche incentivanti di tipo fiscale, ad esempio introducendo nel calcolo dell'ISEE il quoziente familiare ed escludendo dallo stesso il valore della prima casa per i nuclei familiari più deboli. D'altra parte, nel delicato equilibrio tra necessaria ristrutturazione dei conti pubblici e stimolo alla crescita, non possiamo trascurare la parte propulsiva di questo DEF. L'aumento degli investimenti si inscrive in una tendenza positiva che vede il nostro Paese riattivarsi: l'Italia è prima in Europa per l'utilizzo dei fondi del piano Juncker, sfruttando un finanziamento pari a 1,7 miliardi di euro per 29 iniziative e progetti infrastrutturali. Secondo le stime, considerando il cosiddetto effetto leva, potranno essere attivati investimenti pari a circa 12 miliardi e creati circa 3.200 nuovi posti di lavoro. Inoltre, il *masterplan* per il Mezzogiorno, del primo patto - dei quindici totali necessari - per rilanciare il Sud, combinando sia risorse nazionali che europee. fatto cenno al tema trasversale delle infrastrutture. Si tratta di un capitolo che dovrà necessariamente includere la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, che rappresenterà il culmine di un lungo processo volto a concretizzare l'impegno preso dal Governo in merito al completo superamento del *gap* infrastrutturale che separa il Sud dal resto del nostro Paese. Infine, è positiva l'enfasi posta sull'utilizzo completo dei fondi UE della passata programmazione 2007-2013, che ha consentito all'Italia di sfruttare appieno tutto le possibilità di sviluppo offerte dall'Unione e troppe volte andate perdute per nostre mancanze. Il Paese sta dimostrando anche alle parti più intransigenti dell'Unione europea come l'impegno riformatore italiano sia fondato su progetti solidi e stia portando i primi risultati: la riforma del lavoro, i provvedimenti di ristrutturazione del sistema bancario a tutela dei cittadini, la riforma della scuola sono soltanto alcuni dei primi punti messi a segno. La pubblica amministrazione, così come il settore della giustizia, proprio in questi mesi sono oggetto di un processo di profonda innovazione, necessaria per ottimizzare le risorse ed i servizi per i cittadini. In conclusione, il 2016 deve rappresentare lo stimolo per continuare con più convinzione sulla via dello sviluppo ormai intrapresa. Io vorrei ringraziare il Governo e, se mi permette, anche la maggioranza, perché in questo momento di grande difficoltà

prudenza, determinazione e consapevolezza, innovazione e ponderatezza. Pertanto non possiamo che votare convintamente a favore di questo provvedimento.

sui dati dell'ISTAT l'ha già fatta il TG1, perché il direttore Renzi ha già impartito l'ordine, dalle 13,30 alle 17, di dare l'altra menzogna del giorno, cioè che le tasse sulle imprese sono diminuite dell'11 per cento (adesso sembrano Parliamo in termini di aliquote: dal 2014 al 2016 il combinato disposto IRAP-IRES è diminuito di 0,3 punti, dal 33,1 al 32,8

piccoli, come sempre, rimangono fuori. Ho ricevuto dal *premier* Renzi una risposta idiota, perché quell'idiota del *Premier* - me lo consenta - mi ha detto che gli 80 euro a Marchionne allora: non solo ha le visioni, perché vede gufi ovunque, ma invece - guardate, non sono tipa da parlare in questo modo - è lui che porta iella. Addirittura viviamo anche di meno da quando c'è lui. Nel DEF sicuramente qualcosa scritto nero su bianco c'è

di spesa sanitaria sul PIL è la più bassa in Europa e ancora diminuisce, perché nelle vostre strabilianti previsioni il PIL dovrebbe aumentare del 2,8 per cento e la spesa sanitaria solo dell'1,5 per cento. Invece di mostrare tutta questa arroganza con il popolo italiano, con chi chiede chiede finalmente un po' di riguardo e di cura, perché sta rimanendo sempre più indietro, allora perché non la utilizzate magari con il presidente della Bundesbank, che vi ha trattato come degli sciampisti (con tutto il rispetto per le sciampiste), perché vi ha detto: «voi non potete fare le politiche fiscali, io con voi non voglio fare nulla»? Ma chi lo ha nominato, chi lo ha eletto qui in Italia per venirci a dire che cosa dobbiamo fare? Ma perché non pensa lui alla Deutsche Bank, ai 75.000 miliardi di derivati, di cui 34 sono già spazzatura? Perché non pensa a casa sua? Perché noi abbiamo un Governo di pagliacci, abbiamo un Governo che parla di fumetti, che parla di gufi e che non parla di cose serie. Ci dice che l'occupazione sta aumentando. Ma dico, i dati dell'ISTAT, quelli di febbraio, che dicono che gli occupati sono diminuiti del 33 per cento ce li siamo mangiati? Il TG1 perché perché non li ha ricordati? Il direttore del TG1, anzi del "PD1", non lo dice. E poi leggiamo che nelle risoluzioni del Partito democratico c'è il *masterplan* per il Sud. Ma chi volete prendere in giro? Lo state saccheggiando il Sud! Con la decontribuzione avete creato un buco nei conti dell'INPS, perché favorendo le trasformazioni avete fatto sì che le grandi imprese, i giovani Marchionne, quelli che corrono veloci tanto c'è il Governo che elargisce, hanno trasformato i contratti, tanto poi tra tre anni te li mandano a casa, avendo abolito l'articolo 18 con il contratto a tutele crescenti. Ma avete fatto in modo che chi pagava prima dei contributi ora non li paga. A fronte dello stesso lavoratore non abbiamo più i contributi, e imprese, nei cui confronti adesso vantate di avere più fiducia perché dovrebbero pagare meno tasse, in realtà sono passate da 8.000 euro di sgravi a 3.250 per dipendente assunto. Ma a fronte di questo avete eliminato la legge n. 407 del 1990 che favoriva le nuove assunzioni, soprattutto per le imprese artigiane su tutto il territorio il territorio nazionale, non solo per il Sud. Mentite quando dite questo e costava meno di un miliardo. Questo favorino a Marchionne invece ne costa 12 alla fiscalità generale e alle tasche degli italiani.

potremmo recuperare circa 5 miliardi, che dovete usare per disinnescare le clausole di salvaguardia per bloccare voi stessi perché voi le avete messe, i vostri Governi, compreso quello di Renzi, per la marchetta elettorale degli 80 euro per le europee.

Noi non vogliamo il debito per questo. Noi il debito produttivo e lo scostamento vero lo faremo davvero

abbassando le tasse a chi questo Paese lo mantiene. Parlate sempre di evasione e di elusione fiscale; andate nelle banche, nelle assicurazioni, dal padre della Boschi e di Renzi che faceva affari con il padre della Boschi. Di questo dovete parlare. Noi dovremmo dare lo scostamento per fare poi i fondi per aiutare le banche e per poi non restituire neanche il maltolto a chi è stato truffato dal padre del Ministro delle riforme?

poi. Per le altre invece, con la detrazione coniuge a carico, come andrà a finire? Nella delega del *jobs act* l'avete messo che andrete a revisionare quella detrazione. L'avete scritto voi; ve lo siete approvato voi il *jobs act*, mica noi.

costerebbe soltanto 200 milioni, ma voi avete bisogno di recuperare ben 15 miliardi. Allora, la ciccia dove sta? Nella detrazione al lavoro dipendente, nella detrazione per i pensionati e nella detrazione per i familiari a carico. Ditelo questo agli italiani. Andate in televisione e parlate chiaro. Quando andate in televisione a dare sempre dei matti al Movimento 5 Stelle, che accusate perché dice sempre di no, dite anche il perché.

replica ma solo di sentire una propaganda e poi il cittadino si sente quasi in colpa di essere ancora povero. Noi avevamo presentato una Risoluzione che eravamo certi non sarebbe stata accettata e approvata. Abbiamo affidato a questo intervento una preghiera al Presidente del Senato

per quanto riguarda le spese sociali. Vogliamo discuterne? Io vi voglio sentire dire: sì o no. Lo dovete fare in faccia agli italiani. Con questa dichiarazione di voto noi votiamo no a questo DEF e alla relazione per lo scostamento.

però, ci rendiamo conto che mentre la dinamica della macroeconomia internazionale ha aiutato - e non poco - i conti dell'Italia, e l'Italia non è riuscita non è riuscita a monetizzare questi aiuti, a migliorare i suoi parametri di bilancio né a produrre un documento che oggi possa ritenersi esaustivo di un risultato positivo ottenuto,

speranza; di dati attuali che è costretto a riportare in maniera drammatica - lo vedremo - e di dati previsionali che invece vivono, appunto, di ottimismo e di speranza. Tutti gli organismi economici nazionali e internazionali hanno bocciato, senza mezzi termini, l'eccessivo ottimismo di queste previsioni; hanno detto che ci sono rischi insiti sia nella dinamica dell'economia nazionale che in quella dell'economia internazionale; un Governo serio non può non prendere in considerazione questi rischi e che pertanto alcune previsioni, al di là anche degli stessi *spot* che quotidianamente il *Premier* ci propone - e che non troviamo neanche in gran parte riportati nel contenuto di questo documento - non dovrebbero avere luogo per evitare non solo di creare aspettative ma anche per evitare che poi, sull'onda delle aspettative, si realizzino veramente alcuni interventi che peggiorerebbero di gran lunga i nostri conti. Purtroppo per il Governo, i dati di questo primo trimestre del 2016 certificano l'assoluta inadeguatezza delle previsioni e soprattutto delle politiche messe in atto da questo Governo. ai dati sull'occupazione, a quelli sugli investimenti, sul settore creditizio, sulle esportazioni: abbiamo avuto un crollo delle esportazioni. Tutti i dati ci dicono che questo crollo è dovuto principalmente alla chiusura del mercato della Russia, oggetto di incredibili sanzioni da parte dell'Unione europea, e noi continuiamo ad andare in Europa a chiedere l'allargamento

Continuiamo ad alimentare una spesa pubblica che non diminuisce. Mi dispiace dovere entrare in contraddittorio con l'ottimo relatore e con il vice ministro Morando, che ringrazio per la collaborazione che hanno prestato alla 5a Commissione, così come approfitto per ringraziare i senatori Mandelli, Ceroni, Zuffada e Gibiino che sono intervenuti questa mattina esponendo larga parte delle motivazioni che ci portano a considerare questo documento assolutamente inutile e vorrei dire pericoloso. In una sola cosa do ragione al senatore Gualdani: ci vuole proprio coraggio, senatore Gualdani, a presentare questo tipo di documento al Parlamento e soprattutto alla Nazione. La spesa pubblica non diminuisce perché noi guardiamo al valore assoluto; non possiamo guardare al valore relativo, in considerazione di un PIL la cui crescita è prevista e non è reale. Non diminuisce la pressione fiscale. Nella noterella di rettifica che il Governo ci ha trasmesso si è proprio capito che, anche al di là della buona volontà di dare un dato positivo, alla fine la pressione fiscale è diminuita dello 0,1 per cento. Uno 0,1 di pressione fiscale non compensa ciò che gli italiani pagano sotto forma ufficialmente diversa dalla pressione fiscale, ma che pressione tributaria sempre è. Mi riferisco alle tariffe sui servizi degli enti locali: abbiamo avuto un incremento del 20 per cento medio sul territorio nazionale delle tariffe sui rifiuti e sul servizio idrico, che passano per tariffe, ma che in realtà cari colleghi, sono nelle bollette in realtà cari colleghi, sono nelle bollette che ogni giorno arrivano nelle case dei cittadini e che determinano un aumento della spesa verso il settore pubblico. Al cittadino poco interessa che sia tassa, imposta o tariffa: il cittadino sa che aumenta il carico che gli viene chiesto dal settore pubblico

cadde miseramente sotto i colpi di un'elezione contraria; quindi rinviamo: può darsi che sia questo il motivo. Purtroppo, però, il motivo non è questo; il motivo è che non si riesce a diminuire l'incidenza del debito pubblico sul prodotto interno lordo e che tutti i parametri - l'ha detto ieri il Presidente della Bundesbank, della Bundesbank, ma non avevamo bisogno che lo dicesse lui, perché l'abbiamo ripetuto nelle nostre sedi istituzionali in tutti i modi - quella montagna di ghiaccio che ostacola il cammino del Paese, nessuno la vuole considerare. È come se questo Governo fosse sul Titanic che va verso l'*iceberg*, senza voler considerare che questo *iceberg* esiste e che poi purtroppo coinvolgerà nell'affondamento tutto il Paese, continuando a suonare sempre la stessa musica, come le cronache ci riportano: ci riportano: la musica di una manovra espansiva fatta di spesa corrente e non di investimenti. Vorrei dire al senatore Ruvolo: caro amico, la tua immagine salvifica di qualcuno che possa risolvere i problemi i problemi del Mezzogiorno - e della nostra Sicilia, in particolare - dovrebbe passare intanto dinanzi ad un atto concreto, quello della restituzione di quattro miliardi e mezzo di investimenti sottratti al Mezzogiorno con la legge di stabilità per il 2015 a favore della decontribuzione sulle nuove assunzioni da investimenti, quindi da creazione di ricchezza strutturale a spesa corrente effimera, perché tra tre anni quel provvedimento andrà a scadere e - come è stato già detto da qualcuno che mi ha preceduto

che noi non condividiamo, ma che voi avete sempre preso a modello, sosteneva l'utilità dell'investimento pubblico per la crescita. In questo caso, invece, voi volete sostenere l'utilità della spesa corrente pubblica, che dovrebbe andare a favore della crescita. Ma i dati di questi giorni

che giustamente deve annotare le criticità e trasmetterle al Parlamento. Tutti ci dicono che l'economia internazionale potrebbe deteriorarsi e quindi potrebbero non esserci più risparmi sugli interessi del debito pubblico, potrebbe esserci un prezzo del petrolio più alto, potrebbe esserci un dollaro con un rapporto di cambio con l'euro diverso. E noi, dinanzi a tutto questo, non avvertiamo di dover prendere alcuna cautela!

Sì, Presidente. Non sappiamo cosa ci attende nella prossima legge di stabilità mentre vorremmo saperlo prima. Nella nostra proposta di risoluzione avremmo chiesto, ove mai il Governo avesse voluto trarre alcuni spunti, di poter sapere per tempo quali saranno i provvedimenti che si adotteranno con la prossima legge di stabilità. Capisco, perché vivo quotidianamente, la sofferenza del Governo, anche in Commissione; capisco che i panni sono molto stretti, ma purtroppo questi panni si stanno trasformando in stracci che ricoprono a stento il corpo degli italiani.

si sono concentrati con molta efficacia su temi specifici; quindi mi limiterò ad esaminare alcuni aspetti di carattere generale del documento in esame e vorrei cominciare proprio dal contesto internazionale ed europeo,

fino allo scorso anno, una domanda internazionale solida ed invece c'è stato il crollo degli andamenti delle aree emergenti, in particolare il rallentamento forte dell'economia Ci aspettavamo effetti positivi dal deprezzamento nel cambio dell'euro ed invece abbiamo avuto svalutazioni nelle aree emergenti, che hanno in gran parte compensato il dollaro forte. Ci aspettavamo condizioni finanziarie espansive ed in realtà, proprio all'inizio di quest'anno, ci sono stati andamenti dei mercati finanziari, dopo il crollo delle borse, che hanno scosso le attività finanziarie negli Stati Uniti e in Europa. Se non teniamo conto di questi mutamenti è difficile capire le linee di strategia di politica economica contenute nel DEF. Bisogna anche capire che gli andamenti che si stanno determinando a livello internazionale si possono spiegare con il fatto che c'è una carenza di domanda di consumi ed investimenti a livello globale, rispetto alla quale la politica economica dei Governi finora ha fatto molto

Rispetto a questo contesto anche l'Europa ha subito un rallentamento, seppure la crescita è continuata. È vero che le politiche fiscali in Europa sono oggi meno restrittive e che addirittura in Germania si è avviato un relativo aumento della spesa interna, per favorire l'accoglienza dei rifugiati: è certamente qualcosa, ma molto al di sotto di quello che sarebbe necessario. Si può fare molto di più, in particolare cercando maggiori asimmetrie nelle politiche fiscali e soprattutto stimolando una politica di investimenti a livello europeo, andando al di là del pur positivo cosiddetto piano Juncker. Sono investimenti che il nostro Governo richiede da tempo con forza a Bruxelles e che sono in grado di colmare il vuoto che c'è tra una domanda debole e un'offerta in cerca di rilancio. il DEF va letto su questo sfondo, perché su questo sfondo si capisce il quadro tendenziale contenuto nel Documento di economia e finanza ed il quadro programmatico che il Governo si prefigge di raggiungere. Va sottolineata innanzitutto la strategia di politica economica che viene ribadita, giacché ha avuto qualche successo, quella di mettere la crescita al centro, come obiettivo da perseguire e guardare al risanamento della finanza pubblica come ad un vincolo: è una inversione di tendenza importante che è avvenuta ormai negli ultimi due anni, una strategia che stanno seguendo anche molti altri Paesi europei dopo il fallimento delle politiche tutte incentrate sull'austerità, che

ma va subito aggiunto che viene ribadita una linea di prudenza per quanto riguarda il disavanzo pubblico. Infatti, si ribadisce una diminuzione dal 2,6 del 2016 al 2,3, fino all'1,8 per cento, che rappresenta un *deficit* tendenziale superiore a quello previsto, ma che è giustificato dalla necessità di sostenere il percorso dell'economia;

riteniamo soddisfatti di questa dinamica di crescita. Vogliamo fare di più ed è necessario fare di più, anzitutto cercando di stimolare i fattori esterni cui ho fatto riferimento

penalizzano la nostra capacità di crescita: si chiamano bassa produttività, specializzazione produttiva non adeguata a un grande cambiamento in atto a livello internazionale ed europeo e anche una struttura di impresa ancora troppo frammentata.

Ciò significa utilizzare al meglio tutti gli spazi fiscali a disposizione, tenuto conto dei vincoli europei, con i provvedimenti che sono stati già

indirizzato al rafforzamento della capacità di crescita della nostra economia che - è giusto ricordarlo - va stimolata nel suo complesso e soprattutto per quanto riguarda il nostro Mezzogiorno. Con riferimento a questi spazi fiscali disponibili, nel DEF sono contenute delle critiche approfondite e delle proposte motivate per quanto riguarda la modifica delle regole del Patto di stabilità e crescita oggi vigente a livello europeo. le regole europee sono diventate troppo complesse da gestire e spesso sono incomprensibili e in qualche modo anche poco trasparenti.

Come chiede il nostro Governo, l'intento è quello di ridurre gli indicatori e focalizzarci su quelli che sono in grado di essere meglio gestiti. ad esempio, all'evoluzione della spesa pubblica che ci permetterebbe di superare quelle discutibili procedure con cui si calcolano sia il prodotto potenziale, sia il *deficit* strutturale.

che siano praticabili perché noi, come gli altri Paesi dell'area euro, ne abbiamo bisogno. Ma vogliamo appunto regole più facili da rispettare e soprattutto da spiegare all'opinione pubblica. i lavori di revisione sono appena cominciati; richiederanno tempo e non sappiamo nemmeno quali risultati produrranno. Naturalmente è augurabile un esito positivo perché aprirebbe spazi di manovra di cui per primo il nostro Paese potrebbe beneficiare ai fini del rilancio degli investimenti e della crescita, di cui ho parlato in qualche modo prima e che sono poi obiettivi ribaditi e contenuti in questo documento. È per queste ragioni, onorevoli colleghe e colleghi, che ribadisco l'adesione e il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico al DEF e alle proposte di risoluzione che sono state presentate dai

Avverto che per tale deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Pertanto, la votazione della proposta di risoluzione avrà luogo mediante procedimento elettronico con scrutinio simultaneo.

che tratteggia un Paese fondamentalmente diviso. Ho già avuto modo di sottolineare come esista una questione meridionale dentro la questione meridionale, che riguarda l'istruzione e la formazione nelle Regioni meridionali: diritto allo studio, povertà educativa, numero di immatricolazioni nelle università, numero di laureati, numero di studenti che hanno delle borse di studio. Ebbene, quello che ci vuole è un vero e proprio piano Marshall per l'istruzione e l'alta formazione nelle Regioni del Mezzogiorno. Nelle lacunose numerose pagine del *masterplan* sul Mezzogiorno che troviamo nel DEF non si trova nessun accenno a questa gravissima questione. Ecco che il mio emendamento 5.3, nelle linee generali, mira ad introdurre proprio le fondamenta di questo che ho chiamato un vero e proprio piano Marshall, prevedendo delle azioni mirate sulle Regioni meridionali a sostegno dell'istruzione e dell'alta formazione, delle università, degli enti di ricerca, degli studenti e dei ricercatori che lavorano in queste istituzioni di ricerca delle Regioni meridionali. L'emendamento 5.16, che colgo l'occasione per illustrare, signor Presidente, prevede invece delle misure prevede invece delle misure molto più puntuali, che definiscono nel dettaglio cosa deve riguardare questo piano di interventi, in particolare un piano di assunzioni per le università e per gli enti di ricerca a livello nazionale, che preveda delle quote riservate, ancora una volta, per le università e gli enti di ricerca nelle Regioni meridionali. Se dobbiamo riequilibrare il Paese, infatti, è chiaro che dobbiamo prevedere delle misure apposite e delle quote dedicate per le istituzioni che operano nelle Regioni del Mezzogiorno d'Italia. [**Presidenza

Signora Presidente, tutto questo Documento di cui si discute in sostanza stabilisce come allocare risorse e dove recuperarle. Abbiamo sentito tanti interventi e molta preoccupazione per il fatto che c'è sempre il rischio che scattino le clausole di salvaguardia, ogni contribuente vorrebbero dire una mazzata sotto il profilo economico. Propongo all'Assemblea una cosa che non ha nessun costo e non va a toccare i diritti di nessuno. Parliamo della nuova ASPI, cioè dell'indennità di disoccupazione, dell'indennità di disoccupazione, che ha un doppio senso, una doppia funzione. Innanzitutto, consente a chi perde un lavoro o comunque a chi ha un lavoro stagionale (i due settori più toccati sono l'agricoltura e il turismo, che per ovvie ragioni hanno natura altalenante)

Cosa succede però se questo denaro esce dal Paese? Parliamo dei lavoratori stranieri che lavorano per un periodo, dopodiché, poiché non ci sono controlli, tornano a casa propria.

spesa di una famiglia italiana. Noi non tocchiamo i diritti di nessuno: queste indennità possono continuamente essere erogate a una condizione,

i criteri di erogazione; l'indennità non deve essere erogata *una tantum*, dopodiché il cittadino torna a casa sua e chissà se tornerà in Italia, ma deve essere erogata sistematicamente e ciclicamente ogni mese. Quel cittadino, quel lavoratore deve rimanere in Italia, mensilmente deve andare a ritirare ciò che gli spetta, metterà una firma e a questo punto sappiamo che quel sussidio serve per far vivere una famiglia

*relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, in alcuni casi perché esprimono con maggiori e diversi dettagli contenuti già della risoluzione, e in altri casi perché non accoglibili nell'indirizzo della risoluzione.

cioè che la famiglia del lavoratore che ha maturato questo diritto lo debba ritirare mensilmente previa firma; ciò comporterà il fatto che la famiglia spenderà questo reddito in Italia. Se non vogliamo nemmeno questo, secondo me non facciamo neanche il bene del nostro Paese.

testualmente -«rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima contenuta nei prodotti agroalimentari, soprattutto a tutela delle produzioni del comparto lattiero-caseario, al fine di garantire la massima trasparenza, la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera». Cosa c'è di più facile nel dire di sì? Trovate una giustificazione per dire di no.

Presidente, ho voluto ricordare in questo mio intervento - questa non è solo la mia volontà, ma è di tanti democratici, di tanti uomini di sinistra, di tanti sardi - l'anniversario della morte di Antonio Gramsci

bisognava impedire a quel cervello di pensare. E, invece, siamo di fronte a un miracolo perché Antonio Gramsci, in una condizione veramente

Tutti noi ricordiamo il concetto di egemonia con il quale i potenti

opporsi positivamente per creare una società più giusta, più democratica e più a misura dei bisogni dell'uomo. Penso che noi tutti dobbiamo a Gramsci questa capacità di elaborazione, questo pensiero così diffuso. La dobbiamo a un sardo - fatemelo dire - che nasce in un paese della Marmilla, una parte depressa della Sardegna, e che senza mezzi studia con fatica per una tubercolosi ossea che lo farà soffrire per tutta la sua esistenza. Antonio Gramsci, nato in un paese di una parte povera del mondo, in una periferia, è diventato uno dei cervelli più nobili, riconosciuti e apprezzati

le potenzialità che nascono in tutto il mondo, anche nelle zone più sofferenti, vengano portate al massimo della loro espressione. *(Applausi.

vorrei segnalare all'Aula che Messina è nuovamente senza acqua. L'approvvigionamento di questa città dipende da un acquedotto di circa 70 chilometri.

Da quanto mi risulta, il punto in cui ha ceduto non era stato segnalato tra quelle criticità. Il problema è che tutto l'acquedotto è ammalorato e che Messina, che è una città capoluogo di Provincia, è sottoposta continuamente a questo tipo di problema.

l'acquedotto in un punto e si rompe in quello immediatamente successivo, e questa è la situazione - voglio segnalare al Governo il problema. Dai conti fatti, rimettere in sesto il sistema di approvvigionamento idrico della Città di Messina costerebbe 6 milioni,

per quanto mi risulta, oltre al disagio forte dei cittadini non sono sorti problemi di tipo sanitario, ma è inammissibile che nel ventunesimo

che non è la sola in Sicilia, che si ritrova in continuazione di fronte alla mancanza di acqua corrente necessaria ai bisogni quotidiani dei suoi cittadini.